Onorevoli colleghi, ricorreva ieri il 35° anniversario dell'attentato al Tempio maggiore di Roma del 9 ottobre 1982, considerato il più sanguinoso attacco antisemita verificatosi in Italia nel corso del secondo Dopoguerra. Il vile atto criminale fu perpetrato nel cuore della Capitale nelle stesse strade che anni prima, il 16 ottobre del 1943, avevano assistito alla vergogna della deportazione degli ebrei romani nel campo di concentramento di Auschwitz. Il 9 ottobre del 1982 era un sabato, tradizionale giornata dello Shabbat, che coincideva con le celebrazioni legate alla festa delle capanne. Non era stato organizzato alcun servizio di sicurezza fuori dal Tempio. Poco prima di mezzogiorno le famiglie cominciarono a uscire, quando la barbarie assassina si scatenò per circa cinque interminabili minuti, con il lancio di bombe a mano e una serie di raffiche di mitra sparate sulla folla. La cieca e feroce violenza terroristica colpisce sempre i cittadini innocenti: in quell'occasione, l'unica vittima dell'ignobile attentato fu un inerme bambino di soli due anni, Stefano Gaj Taché, mortalmente colpito dalla scheggia di una bomba a mano. Una quarantina di persone vennero ferite e fra loro anche i genitori della piccola vittima e il fratello Marco Gadiel, che all'epoca aveva quattro anni, che oggi sono qui con noi. Li saluto con affetto.

Per riprendere le parole del Presidente della Repubblica nel discorso di insediamento del 3 febbraio 2015, Stefano Gaj Taché. «Era un nostro bambino, un bambino italiano», suo malgrado tristemente assurto a simbolo del prezzo pagato dal nostro Paese sull'altare dell'odio e dell'intolleranza. L'anniversario del tragico attentato non può non indurre le istituzioni e cittadini a una serie di riflessioni e a un rigoroso esame di coscienza collettivo. L'attacco al Tempio maggiore di Roma risveglia in noi l'incubo del mostro antisemita, i cui rigurgiti, seppur isolati, purtroppo persistono ancora nella nostra società e, più in generale, nel mondo occidentale. Riemergono le assonanze con gli atti terroristici che in tempi recenti hanno funestato diverse città d'Europa e di altri Continenti. Ad accomunarli è il medesimo sentimento di odio e la volontà di annientamento del nemico, il tutto ammantato dall'utilizzo della violenza come arma di lotta politica e dall'esaltazione del fanatismo religioso. La ricorrenza di ieri rappresenta quindi un monito a tutti noi per riaffermare il primato dei valori della libertà, della pacifica convivenza tra popoli e religioni, della tutela dei diritti di tutte le minoranze, oltre che del fermo rifiuto di qualunque tentativo volto a giustificare la violenza quale strumento di affermazione politica o di prevaricazione di un credo religioso. anni dall'attentato al Tempio maggiore di Roma, appare doveroso rinnovare, a nome dell'intero Senato della Repubblica, un sentito e profondo sentimento di cordoglio alla famiglia del piccolo Stefano, vittima innocente della ferocia terroristica, e rivolgere un abbraccio e un pensiero di stretta vicinanza a tutte le persone colpite, ai loro cari, alla comunità ebraica, rappresentata oggi in Senato dalla presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni da una delegazione della comunità ebraica di Roma guidata dalla presidente Ruth Dureghello, che sono qui con noi in tribuna, nonché un saluto e un abbraccio ai cittadini di Roma. Invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

del giorno reca la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Cosenza. Con ricorso depositato l'8 febbraio 2017, il tribunale ordinario di Cosenza - seconda sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta antimeridiana del 16 settembre 2015, ha dichiarato l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Antonio Gentile, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi allo stesso tribunale di Cosenza - seconda sezione civile Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 7 giugno 2017, n. 155, depositata in cancelleria il successivo 4 luglio. Nella seduta del 27 settembre 2017, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

colleghi, l'oggetto su cui l'Assemblea è chiamata a esprimersi oggi riguarda esclusivamente - ribadisco: esclusivamente l'eventualità di una costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto d'attribuzione sollevato, a nostro avviso, in maniera del tutto legittima, dal tribunale di Cosenza in relazione a un procedimento civile riguardante il senatore Antonio Gentile. Com'è noto, infatti, l'Assemblea del Senato, in data 16 settembre 2015, ha approvato la proposta formulata dalla Giunta di dichiarare insindacabili le dichiarazioni del senatore Gentile stesso. Per le ragioni già ampiamente esposte in quella sede, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha votato in senso assolutamente contrario, ritenendo assolutamente doveroso il procedimento civile a carico del senatore Gentile, giudicabile dalla magistratura ordinaria come tutti gli altri cittadini italiani. Ribadisco: come tutti gli altri cittadini italiani. L'effetto diretto della costituzione in giudizio del Senato dinanzi a tale procedimento non può che essere quello di nominare un avvocato, guarda caso con un ulteriore costo per i contribuenti, che avrà il mandato di sostenere dinanzi alla Corte costituzionale le medesime tesi, secondo noi - lo ribadiamo - errate, già sostenute dall'Assemblea del Senato nel momento in cui ha dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Antonio Gentile. L'eventuale mancata costituzione in giudizio della parte resistente non comporta, tuttavia, l'estinzione del giudizio, che quindi si potrà ugualmente svolgere anche senza la necessità che l'apporto argomentativo del Senato abbia a riprodursi, essendo già stato abbondantemente espresso nelle deliberazioni sia della Giunta che dell'Assemblea del 2015. Siamo di fronte, pertanto, a un mero aspetto di dialettica processuale che, essendo il *thema decidendum* ben circoscritto del ricorso e già sviluppato nell'atto promosso dal tribunale, nulla può aggiungere e nulla può togliere all'accoglimento nel merito della questione sollevata

di un appesantimento rituale determinato solo da una consolidata prassi e, comunque - lasciatemelo dire - oneroso,

che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha reiteratamente proposto di sottrarre alle Camere la possibilità di giudicare i suoi stessi membri, assegnando tale compito in via esclusiva alla Corte costituzionale. Questo, e soltanto questo, supererebbe il vetusto e iniquo principio secondo cui chi appartiene alla casta dei parlamentari può giudicare se stesso, determinando reiterate aberrazioni giuridiche. È questa l'autodichia, che sottrae alla giurisdizione ordinaria il parlamentare. Per i motivi esposti, pertanto, il Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle voterà contro la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in oggetto.

non si può rinnovare inutilmente ciò che rappresenterebbe, allo stesso modo, un onere per il contribuente. Che il procedimento ormai vada avanti, visto che dovrà andare avanti e quanto meno risparmiamo i soldi dei cittadini italiani.

per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Cosenza - seconda sezione civile. **È approvata.**

Noi stiamo annacquando l'Olocausto in altre migliaia di fattispecie che riguardano crimini di guerra, genocidi e crimini contro l'umanità, quindi mettiamo sullo stesso piano un singolo episodio di guerra, che può essere costato la vita

la pena sostituisce la multa o i diciotto mesi di carcere con un minimo di due anni ed un massimo di sei anni di pena. E questa tegola a chi capita in testa? Al malcapitato che pubblica una "grave minimizzazione" di migliaia di fatti, quelli indicati nei famosi articoli della Corte internazionale, anche se non c'è una sentenza passata in giudicato. Basta che sia nell'elenco. Ricordo al collega Malan e agli altri colleghi che hanno fatto disinformazione che qui non si parla di apologia né di incitamento dell'odio, si parla semplicemente di uno storico o di un giornalista che scriva un articolo o pubblichi un libro

può portare all'incriminazione. Ma che cosa è la "grave minimizzazione"? Colleghi, qualcuno di voi mi sa dire cosa vuol dire "grave minimizzazione" di un fatto e non la negazione dello stesso? E mi sa dire come sia possibile, in un Paese civile e democratico, introdurre pene fino a sei anni per reati che sono soltanto di opinione, come una ricostruzione che lo storico o il

storico, giurista e uomo di cultura, ricordando che un anno fa questo Senato ha stralciato la minimizzazione perché è una aberrazione giuridica e la Commissione giustizia ha portato alla Commissione referente un parere in cui si diceva che eravamo in piena illegalità. La Corte costituzionale ha bollato tali norme penali come non rispondenti al principio di tassatività e al principio di legalità. Noi stiamo riempiendo il codice penale di norme talmente vaste che poi sarà il processo a stabilire se nei limiti e negli ambiti della minimizzazione il reato è stato provocato o no, ma intanto la persona viene denunciata la persona viene denunciata e si trova sotto processo per una fattispecie penale che non soltanto è assolutamente indeterminata, ma è anche una lesione dei principi fondamentali della libertà di ricerca storica, è una lesione ai principi fondamentali della possibilità di indagare, di verificare e di fare giornalismo. Non c'è apologia, non c'è istigazione all'odio, c'è solo un'opinione che interpreta un fatto in maniera diversa. Ricordate, colleghi, per quanti decenni le fosse di Katyn furono attribuite alla barbarie nazista? Poi, la ricerca storica ha portato a stabilire che quelle decine di migliaia di ufficiali furono eliminati da Stalin e dall'Unione sovietica. E allora, che cosa facciamo? Dobbiamo lasciar passare alla storia un fatto come assolutamente ingiustificato perché in un primo tempo l'attribuzione era stata di un certo tipo? Ma la ricerca storica, allora, a cosa serve? Mi richiamo anche alla discussione di questa mattina: alle statue di Cristoforo Colombo, alla rilettura del passato, a questo fanatismo ideologico che vuole cancellare ogni forma di dissenso rispetto a un'interpretazione storica che può essere in divenire, ma che deve anche tener conto delle condizioni nelle quali sono avvenuti gli avvenimenti. All'epoca dell'antica Roma c'era una certa mentalità, nel Medioevo ce n'era un'altra, nel Risorgimento un'altra perché se no rileggiamo la guerra al brigantaggio fatta dai piemontesi nelle Regioni meridionali e magari anche quelli erano crimini di guerra. Può darsi, non so se se fossero o meno crimini di guerra, ma certamente definire questo viene demandato alla ricerca storica e non al fatto che un tribunale arrivi a dire che un soggetto sta minimizzando quello che qualcuno può pensare sia stato un genocidio.

L'Europa ce lo aveva chiesto anche l'anno scorso: c'è un'infrazione, andremo a spiegare che il nostro ordinamento non lo consente. Poi, colleghi, io sono filoisraeliano, filoebraico da sempre e qualcuno mi deve spiegare perché noi minacciamo sei anni di carcere carcere per chi difende Israele nel caso in cui un tribunale internazionale o un organismo come l'ONU stabilisca che, con un suo intervento a Gaza, Israele abbia compiuto un crimine di guerra.

non potrà più esprimere un'opinione di questo tipo, in Germania vengono eletti decine e decine di deputati neonazisti, il capo del partito e il vice presidente negano totalmente l'Olocausto, e nessuno dice niente. Vorrei capire in che razza di mondo viviamo e l'Europa che cosa sta facendo: perseguita chi va a fare una ricerca storica su un avvenimento dei Balcani e poi non dice nulla davanti a un Gruppo parlamentare in Germania, nato proprio sulla base di considerazioni antisemite e di rivisitazione e negazione dell'Olocausto, che arriva in Parlamento e anzi guadagna dei voti? Qualcuno di voi non è sfiorato dal pensiero che queste norme, lungi dall'aiutare a creare una cultura di tolleranza, di comprensione, di condanna di quello che è stato il passato, proiettandolo verso il futuro, creano soltanto sconcerto?

L'ho detto scherzando, mica tanto, perché cos'è il reato di xenofobia? Una discussione sulla migrazione o sui flussi migratori o sulla necessità di regolarli piuttosto che sulla necessità di tener conto anche di fattori religiosi è forse xenofobia?

Per fortuna, i giornali se ne sono accorti. Stamattina qualche autorevole settimanale e quotidiano hanno posto il problema. Ricordo ancora che tutti gli storici interpellati, non solo quelli presenti in quest'Aula, da Flores

contrari a questa norma. L'hanno scritto sul «Corriere della Sera», su «La Repubblica», su «La Stampa»: la considerano una minaccia alla libertà di ricerca. A tutte queste motivazioni che noi portiamo che cosa si risponde? Semplicemente che

come indicato ovviamente nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie, quali le indicazioni del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in chilogrammi, il nome o la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine, nel caso di provenienza da un Paese terzo, che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento. Ora, non è una questione di vita o di morte, sia chiaro, e non è una questione decisiva per il contenuto, però è un abbassamento di tutele che, a mio avviso, può essere semplicemente eliminato con la soppressione del comma 5, come prevede l'emendamento 12.1 a mia prima firma, oppure - illustro anche l'emendamento 12.3

Ho riflettuto a lungo prima di presentare l'emendamento e non riesco a trovare una ragione valida se non una attenuazione che risponde, a mio avviso, ad altre logiche e ad altri interessi che non meritano tutela, visti gli sforzi che quest'Assemblea,

Come il collega già ha indicato, risulta difficile comprendere la *ratio* per la quale il Governo non accetti questo tipo di modifica. «soltanto» esclude una tutela dei consumatori, perché limita l'indicazione in etichetta soltanto al documento di accompagnamento per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie. Giova ricordare che il comma 5 recita: «Possono essere riportate soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 3, lettere *b)*, numero

terzo. Abbiamo purtroppo assistito prima alla chiusura del confronto con un voto tranciante per quanto riguarda l'articolo 5. l'articolo 5. Nel confronto svoltosi prima dell'inizio della seduta abbiamo saputo dal Governo che non c'è intenzione di apportare modifiche al provvedimento per non ritornare alla Camera.

da sempre ci impegniamo nel promuovere una politica che renda consapevole il consumatore in merito al prodotto da acquistare. Qualsiasi indicazione che attenua questo diritto del consumatore, ovvero che facilita l'ingresso sul mercato di prodotti

Scegliete se toglierlo; scegliete se, come indicato dall'emendamento del collega Ruta, inserire «anche» al posto di «soltanto», ma prendete una posizione. Il problema non è nel tornare alla Camera con un voto veloce che questo provvedimento viene rallentato, ma è la qualità, la bontà, di questa legge che, così come è fatta, onestamente ci lascia molti perplessi.

Ci saranno dei decreti da fare e un successivo passaggio normativo. Prendetevi un impegno,

in effetti, si potrebbe pensare a una trasformazione in un ordine del giorno unitario, in riferimento al comma 5 dell'articolo 12, per invitare il Governo a valutare la possibilità di sostituire la parola "soltanto" con la parola "anche" e quindi andare nella direzione auspicata dai presentatori degli emendamenti rispetto all'obbligatorietà di riportare,

credo che la proposta della relatrice di trasformare gli emendamenti 12.2 e 12.3 in un ordine del giorno raggiunga l'obiettivo perseguito dai due proponenti. Pertanto il Governo è favorevole alla proposta della relatrice.

L'ordine del giorno assorbe il concetto della soppressione, in quanto impegna il Governo in una certa direzione. I tre emendamenti sono quindi assorbiti dall'ordine del giorno, che poi potremo

concordo con la posizione assunta dal senatore Martelli, perché è evidente che la trasformazione degli emendamenti nell'ordine del giorno è riferibile all'emendamento 12.2, a

Mi scusi senatore Calderoli, credo che l'interpretazione degli emendamenti e la loro trasfusione in un ordine del giorno appartenga al relatore.

procederemo alla sua votazione. Non credo ci sia una gran difficoltà. Quello che era stato detto dal presentatore era diverso: pertanto non c'è un'ostilità a questo fatto.

diminuzione della difesa del consumatore, ma vorrei dire anche del piccolo produttore. Non per nulla, gli emendamenti vengono prevalentemente da componenti della Commissione agricoltura, cioè da coloro che, nell'ambito delle Commissioni permanenti, sono preposti a difendere i diritti e le prerogative dei nostri produttori.

un'ulteriore delegittimazione delle fonti normative primarie. Se la fonte normativa primaria rimane la legge, non vi può essere alcun regolamento, per quanto ci si arrampichi sugli specchi, che possa introdurre una modalità comportamentale diversa.

assumere ogni iniziativa utile affinché, alla luce dell'esito della procedura EU/Pilot in oggetto, la classificazione di sfalci e potature sia coerente con la vigente legislazione europea.

ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori». Quando ne abbiamo discusso in Commissione, ci siamo trovati d'accordo

chiarezza e di conoscenza per i cittadini in merito ai dati di monitoraggio. Per tale ragioni voteremo a favore dell'emendamento.

contrario del Governo non c'entra nulla con la necessità di evitare una terza lettura, posto che il Governo ritiene che la terza lettura sia inutile e che costerà probabilmente l'apertura di alcune procedure

la ragione del parere contrario del Governo, che non è legata alla necessità di evitare una terza lettura, altrimenti, dovendo fare una terza lettura, sarebbe facile per il Governo dare parere favorevole anche su questo punto. La ragione per cui il Governo dà parere contrario non è la terza lettura, ma il fatto che ciò che il fatto che ciò che il senatore Candiani richiede è già previsto in quanto gli obblighi concernenti l'accesso del pubblico all'informazione ambientale sono contenuti nell'articolo 78 del codice dell'ambiente. dell'ambiente. Non c'entra nulla con la terza lettura, ma con il fatto che è perfettamente inutile aggiungere una disposizione di legge, quando tutti vogliamo semplificare, a una già prevista all'articolo 78 del codice dell'ambiente, che dispone la pubblicazione del piano di gestione dei bacini idrografici, il quale contiene anche le informazioni relative ai programmi di monitoraggio e ai relativi risultati. Il senatore Candiani lo sa perché ho avuto modo di spiegare questo aspetto anche in Commissione. Confermo

Signora Presidente, rientra nelle mie prerogative di parlamentare esprimere il mio pensiero.

noi parliamo delle autorità di distretto ben sapendo che sono state soppresse le autorità di bacino. Le autorità di distretto, che hanno una funzione gestionale, si trovano in una situazione un po' strana, perché la soppressione delle autorità di bacino, senza aver fatto

Detto questo, ribadisco che la nostra posizione sull'emendamento 16.2 è assolutamente favorevole, perché riteniamo che le cose debbano essere chiare e specifiche. Infine, ribadisco al Governo che se il Parlamento viene accusato di produrre procedure di infrazione, è bene che l'Esecutivo guardi prima in casa propria. Infatti, diverse cose fatte da questo Governo hanno provocato procedure di infrazione. Quindi, ognuno si assuma le proprie responsabilità e il Governo impari a fare il Governo così come noi siamo bravi a fare i parlamentari,

però il tema della procedura europea è reale e non si deve risolvere penalizzando

per gli sfalci e le potature provenienti da attività di manutenzione del verde urbano, costringerebbe tutti i Comuni d'Italia

Chiedo scusa per la mia voce, che oggi non è delle migliori, e forse qualcuno ne può essere contento. Il problema è che reintrodurre la nozione di rifiuto per sfalci e potature del verde urbano significa gravare i Comuni di un onere non indifferente, quindi vorrei pregare il Governo di riflettere sul parere favorevole che viene dato a questo concetto.

i Comuni italiani uscirebbero con le ossa rotte dalla reintroduzione del concetto di rifiuto per quanto riguarda gli sfalci e le potature urbane, che per ora possono essere esitate in maniera molto meno onerosa.

L'ipotesi è di trasformare l'emendamento 22.1 in ordine del giorno per assimilarlo al G22.200, ma cambiando l'impegno, modo seguente: «impegna il Governo a sviluppare, d'intesa con i due rami del Parlamento, modalità uniformi di attuazione degli obblighi d'informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012, così da permettere alle Camere il più informato esercizio della funzione legislativa nelle materie europee, garantendo nel contempo la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti rispetto a soggetti terzi».

Presidente, apprezzo lo sforzo della relatrice, ma onestamente l'ordine del giorno vuole andare proprio nella direzione della massima massima trasparenza della documentazione, e non rispetto a terzi. Stiamo parlando della documentazione a disposizione dei parlamentari, per cui non capisco la confusione che la relatrice sta facendo proponendo la necessaria riservatezza verso terzi rispetto a un ordine del giorno che vuole mettere a disposizione dei parlamentari che compongono la Commissione

per disciplinare la previsione dell'attuazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 4, 14 e 15 della legge n. 234 del 2012. Trattandosi di informazioni contenute in atti riservati, e quindi non provvedimenti legislativi, a Governo e Parlamento, la formulazione riguarda anche la necessaria riservatezza delle informazioni rispetto ai terzi. L'impegno rispetto ai membri della Commissione c'è e si richiede un protocollo che renda modalità uniformi per i due rami del Parlamento.

europei richiede la riservatezza. E, quindi, dobbiamo lavorare, da una parte, per assicurare l'obbligo di riservatezza rispetto al pubblico e, dall'altra parte, per garantire, alla luce degli impegni che abbiamo assunto, la massima informazione possibile ai parlamentari. Ricordo, tra l'altro, Presidente, che il Governo ha proposto alla Camera e al Senato

- l'esigenza di informazioni in una fase di precontenzioso EU Pilot o di contenzioso d'infrazione, nella quale siamo obbligati, in base al regolamento europeo di accesso agli atti, a mantenere la riservatezza.

nelle materie europee, garantendo nel contempo la necessaria riservatezza delle informazioni e dei documenti rispetto ai terzi». Se questa riformulazione, che credo venga incontro alle esigenze della senatrice Montevecchi, verrà accolta, il parere del Governo è favorevole.

Signora Presidente, vorrei richiamare l'attenzione di tutti i colleghi dell'Aula su questo articolo, che riguarda la cosiddetta *data retention*. Nell'articolo 23 il Governo ci propone, in applicazione - secondo il Governo - della direttiva 2017/54, di innalzare il periodo di *data retention* delle telefonate, delle comunicazioni via Internet, degli SMS e delle chiamate (anche senza risposta) a un periodo di sei anni. Tale articolo è stato dichiarato in palese contrasto con la giurisprudenza e la normativa europea dal garante per la protezione della *privacy* Antonello Soro, in una sua intervista che risale a qualche mese fa, quando questo provvedimento è passato alla Camera.

e non assolutamente di comunicazioni elettroniche, di telefonate e SMS. La direttiva ci esorta semplicemente ad adottare sanzioni e misure di contrasto necessarie e a provvedere alle misure di protezione, assistenza e sostegno per le vittime del terrorismo.

Ricordo a quest'Aula che in Europa si tentò, nel 2006, di introdurre una direttiva europea per la *data retention,* che - pensate - a quell'epoca prevedeva la conservazione dei dati per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi. E ripeto ventiquattro mesi, mentre noi qui stiamo parlando di sei anni. E tale direttiva sulla *data retention* è stata dichiarata dalla Corte di giustizia europea

Nell'articolo 24, signora Presidente, il Governo ci propone di aumentare la *data retention* in maniera indiscriminata per un periodo di sei anni. sottolineare che il Governo potrà utilizzare una siffatta schedatura indiscriminata delle comunicazioni dei cittadini italiani non solo per i reati di terrorismo, ma anche per tutto un altro elenco di reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a),* del codice di procedura penale. Quindi, il Governo sta dirittura ampliando le fattispecie per le quali potrà utilizzare una illiberale e indiscriminata raccolta raccolta selvaggia di dati per reati che esulano dalla direttiva europea. Signora Presidente, io richiamo tutti i colleghi di quest'Aula a prendere in altissima considerazione il voto che stiamo esprimendo sull'articolo 24

Signora Presidente, onorevoli colleghi, a settantuno giorni dall'approvazione della legge di delegazione dello scorso 2 agosto ci troviamo a discutere e votare la quinta legge europea. Il provvedimento, *omnibus* per sua stessa è volto a sanare - su indicazione della Corte di giustizia e della stessa Commissione - gli errori della legislazione nazionale. Nello specifico consente di chiudere tre procedure di infrazione, concernenti il fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti; il ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi, in favore dello Stato, in relazione

tre casi EU Pilot in materia di particolari forme ed espressioni di razzismo, xenofobia e negazionismo - sui quali, peraltro, ben conosciamo il dibattito che in questa Assemblea si è scatenato - di agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri dei Paesi dell'Unione europea e di trattamento economico degli ex lettori di lingua straniera in servizio presso le università statali. Altre disposizioni, come sempre accade, sono state inserite successivamente. Il testo, infatti, è stato profondamente modificato dalla Camera dei deputati, che ne ha addirittura raddoppiato il numero degli articoli. Il sottosegretario per le politiche europee Gozi auspicava una discussione del provvedimento approfondita in prima lettura e celere in seconda, in modo da garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa europea. Detto, fatto: sembrerebbe che questo provvedimento debba essere semplicemente vidimato. Tuttavia, vorrei richiamare alcuni punti che credo meritino una riflessione. Da un lato, il Governo sottolinea con orgoglio il numero delle procedure d'infrazione, dal 2014 a oggi, è stato dimezzato: siamo passati da 216 a 65, ed è vero, bene; dall'altro, però, omette di dire che nell'ultimo anno sono state aperte a nostro carico ben otto procedure su argomenti che spaziano dalla concorrenza, alle buste di plastica, alla lotta contro i ritardi di pagamenti transnazionali. A fronte delle tre chiuse ve direi che il saldo non possa essere definito ottimale, perché siamo a più cinque. Inoltre abbiamo aggredito, negli ultimi due anni, le procedure di infrazione più semplici, sorvolando sulle procedure a carico dell'Italia ad esempio - in tema ambientale, in particolare su discariche e rifiuti pericolosi. Non abbiamo ancora provveduto a chiudere le procedure a nostro carico aperte sin dal 2003 che spaziano dall'ILVA di Taranto allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, dalla normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche fino alla costruzione - incredibile, ma vero - di una nuova sede per gli uffici giudiziari nel Comune di Bari. Qualche riflessione vorrei porre anche su alcuni articoli: è stata - ad esempio - persa l'occasione, all'articolo 2, di recepimento della direttiva 2014/26/UE, quella che in astratto consentirebbe la libera scelta dell'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore; una battaglia, questa, condivisa con molti altri colleghi, indipendentemente dallo schieramento e vorrei citarne alcuni: Ichino, Gambaro, Montevecchi, Ceroni fino, naturalmente, al mio presidente di Gruppo, Gaetano Quagliariello. Eppure, il Governo rimane sordo agli appelli, accettando un mero ordine del giorno, svuotato del suo profondo valore, tarpato e reso innocuo, fino a diventare una mera valutazione di opportunità di omologazione alle prescrizioni della commissaria per il digitale Gabriel. Vorrei sapere per quale motivo il Governo preferisce promettere - per tramite del sempre gentilissimo sottosegretario Gozi di inserire la stessa norma, da me proposta come emendamento al provvedimento in esame, nella futura legge di bilancio, invece che provvedere immediatamente a tutelare artisti, interpreti ed esecutori, che ad oggi continuano, per l'incomprensibile ostinazione di qualcuno, a essere costretti per legge ad affidarsi alla gestione esclusiva - e direi medioevale - dei propri diritti da parte del monopolio SIAE. Fortunatamente la discrezionalità dell'Esecutivo ha un limite, quello del voto parlamentare, e noi aspetteremo di vedere la legge di bilancio per capire se *pacta sunt servanda*, ovvero se quanto promesso è un concetto generalmente accettato, o se la maggioranza ne darà una interpretazione diversa. Il disegno di legge in esame interviene anche su un settore che ai nostri rappresentanti al Parlamento europeo, oltre che al Governo, dovrebbe stare a cuore: le eccellenze alimentari. All'articolo 12 si prevedono disposizioni attuative in materia di caseine e caseinati destinati all'alimentazione umana. Sorvolando sulla prima osservazione, e cioè che avremmo dovuto implementare questa direttiva

preferisco concentrarmi su un tema ancor più importante attinente il merito. Non riuscire a difendere le nostre istanze a Bruxelles consentire che i nostri produttori caseari perdano la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali di produzione dei prodotti caseari in favore di regole dettate da chi non possiede il nostro *background* alimentare, significa condannare quelle eccellenze, che dovrebbero essere la punta di diamante della nostra economia, in un contesto di commercio globalizzato. Con tale articolo si vieta la commercializzazione dei prodotti non conformi alla nuova normativa oltre il termine il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Mi chiedo, dunque, se qualcuno degli autori di questa brillante novella normativa abbia una vaga idea del tempo di stagionatura dei prodotti caseari.

Andate a chiedere da 1.000 a 10.000 euro ai nostri allevatori, che ad oggi, nelle Regioni colpite dal sisma, non hanno ancora ottenuto una sistemazione dignitosa *(Applausi del senatore Quagliariello)*. Peccato che abbiate perso, in una sorta di delirio collettivo, il senso della vergogna Se, da un lato, i nostri rappresentanti presso le istituzioni di Bruxelles non riescono a ottenere una specifica regolazione su temi a noi cari, dall'altro lato, c'è da notare che noi stessi siamo costretti - e l'articolo 16 ne è una dimostrazione - ad ammettere che da soli non riusciamo a tutelare le nostre ricchezze. La disposizione di tale articolo è finalizzata a sanare una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI, relative alla non corretta applicazione della direttiva 2009/90/CE, che stabilisce specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. La "rivoluzione copernicana" che introduciamo tramite questo articolo consiste nell'assicurare gli *standard* di qualità e l'intercomparabilità a livello di distretto idrografico dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche e, di conseguenza, dell'effettivo stato chimico dell'ecosistema dei corpi idrici superficiali, in quanto ad oggi, a causa delle molteplici autorità e della burocrazia nel settore, derivanti da anni di legiferazione sul tema senza un organico progetto, non siamo in grado di confrontare i dati di monitoraggio. Il Gruppo di Federazione della Libertà, considerati i pro e i contro, voterà contro il provvedimento in esame, perché, oltre alle aberrazioni dell'articolo 5, non sana realmente le carenze strutturali del Paese e non fa altro ch sfiorare la superficie di un problema più ampio. Rimane, tuttavia, la necessità di recuperare la nostra credibilità nei confronti dei *partner* europei, che passa inevitabilmente attraverso un serio impegno non solo legislativo, ma anche politico, volto a chiudere le procedure di infrazione a nostro carico e un costruttivo confronto con le istituzioni comunitarie sulle regole che non possono considerarsi eque nei confronti dell'Europa mediterranea alla quale noi apparteniamo. Carta moneta di recente prodotta in Francia, aziende d'eccellenza svendute e poi preoccupiamoci dello *ius soli:* tra un po' magari, continuando così, nessuno più sarà così temerario da chiedere la cittadinanza a questo Paese bellissimo, ma sfortunato, e avremo risolto, all'italiana maniera, anche questo difficile problema. colleghi, sottosegretario Gozi, stiamo trattando in seconda lettura un provvedimento scarno, ormai azzoppato, quando in una parte dell'Europa rischia di divampare un incendio. Sul *referendum* della Catalogna di domenica 1° ottobre abbiamo assistito a tante follie, una violenza inaudita da parte della Guardia civile spagnola, ma anche a silenzi imbarazzanti di questa Europa senza autorevolezza.

Tutti abbiamo visto le immagini: militari in tenuta antisommossa che hanno sfondato con la forza seggi elettorali ed esercitato violenza su cittadini, donne, uomini e anziani, calpestandoli, usando manganelli e proiettili di gomma solo perché chiedevano di votare; militari che hanno manganellato i *bomberos* catalani; i vigili del fuoco che facevano scudo ai cittadini scesi in piazza Barcellona; *bomberos* che sono diventati, per quel gesto, degli eroi. Si tratta di violenze che in Spagna rischiano concretamente di riportare indietro l'orologio della storia di oltre quarant'anni, quando vi era la dittatura franchista. È davvero inconcepibile che, dopo quanto è successo, il Parlamento europeo e la Commissione europea tacciano, minimizzino; che il presidente Juncker e la stessa Merkel dicano, con atteggiamento pilatesco, che si tratta di un affare interno allo Stato spagnolo. Ed è davvero inquietante che in Italia ci sia stato qualcuno che ha esaltato il Governo di Madrid, che ha liberato a randellate i seggi elettorali, prendendosela con donne, anziani e bambini. Si conferma che questa non è l'Europa che sognavamo, che disattende persino il Trattato su cui si fonda l'Unione, che all'articolo 2 afferma che l'Unione europea si fonda certamente sui valori del rispetto dello Stato di diritto, ma anche sui valori del rispetto della dignità umana, dei diritti umani, della libertà e della democrazia. In Catalogna, libertà e democrazia sono stati invece violentati e nessuno ha aperto bocca. Nessuno ha garantito questi valori, né ha censurato chi questi valori ha calpestato. L'Europa ha dimostrato, per l'ennesima volta, la sua ipocrisia, così come ripetutamente Bruxelles sta dimostrando con le reiterate sanzioni contro la Russia, perché Putin è considerato non democratico; sanzioni che nuocciono enormemente anche alle nostre imprese. Vergognoso è il silenzio su oltre 800 cittadini manganellati, mandati all'ospedale perché chiedevano il diritto di votare. La violenza non è mai la soluzione: se vince la violenza, è morta la politica. Quello che si sta paventando in Spagna, la più grave crisi del dopo Franco, dovrebbe preoccupare tutti, *in primis* le autorità europee, ma si sa: lì comandano solo i tecnocrati. Madrid ha deciso di mandare a Barcellona l'esercito per gli sviluppi che potrebbero esserci nelle prossime ore e minuti. Il Governo spagnolo ha già iniziato a presidiare obiettivi strategici come l'aeroporto e gli uffici giudiziari. Rajoy ha detto che impedirà l'indipendenza. L'Unione europea dovrebbe battere un colpo e invece fa poco o nulla. Domando: perché due pesi e due misure? Perché nel febbraio 2008, all'indomani della proclamazione dell'indipendenza unilaterale dalla Serbia da parte del Parlamento kosovaro, a Bruxelles è stato convocato subito un Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea, chiamato a prendere posizione su quella questione? L'obiettivo allora era tentare di raggiungere un difficile compromesso tra le diverse posizioni in campo e ricordo che allora, in quell'occasione, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna

per aiutare Madrid e Barcellona al dialogo e trovare un punto di caduta democratico. Diversamente, la situazione potrebbe veramente sfuggire di mano e deflagrare con una *escalation* di disordini e violenza. Mi avvio alle conclusioni, tornando alla legge europea 2017, mentre - ripeto - il governo europeo resta alla finestra rispetto ai gravi fatti della Catalogna. Non condividiamo questo assurdo metodo di normare e omologare il tutto, sopprimendo le specificità, peraltro introducendo cose gravissime, come la norma che, a gamba tesa, amplia il campo di applicazione dell'aggravante del negazionismo, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione, come ha detto bene la settimana scorsa la collega Erika Stefani in discussione generale. Basta introdurre nuove fattispecie di reati di opinione difficilmente dimostrabili. *(Applausi Gravissima poi la censura sul *web*. Inaccettabile dare la facoltà all'Agcom di accogliere l'istanza dell'autore per la tutela dei diritti: un potere che potrà disporre la cancellazione dei contenuti dal *web*. Questa è una censura alla Rete. Attribuire all'Agcom, un'autorità amministrativa, il potere di sequestrare il *web* è allucinante; è esattamente il contrario di quello che prevedono le norme europee, cioè che la competenza deve essere dell'autorità giudiziaria. Sottosegretario Gozi, ma la legge europea non dovrebbe dirimere le controversie con l'Europa? Qui stiamo invece ponendo le condizioni per una nuova procedura d'infrazione. Alla Camera sistemi questa norma, ovviamente se questo procedimento ci arriva. Tutte queste cose non possono che portarci sempre più lontani da un'Europa che non è quella dei popoli, ma sempre più quella delle banche e dei burocrati. Così non va bene; l'Europa deve essere assolutamente cambiata. È per questo motivo che il voto finale del Gruppo della Lega Nord non potrà che essere di assoluta contrarietà su questo provvedimento.

ma un intervento sulla legge europea che stiamo approvando; credo che sia più consono al dibattito dopo gli articoli che abbiamo approvato oggi, perché ritengo che la secessione della Catalogna sia un affare interno della Spagna. Quello in discussione oggi è un provvedimento estremamente rilevante, le cui disposizioni, sebbene molto eterogenee fra loro, si rendono necessarie in funzione di quel processo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello europeo in corso da tempo. Norme come queste sono dunque indispensabili per arrivare a quell'armonizzazione normativa sovranazionale, utile anche a uscire dal circolo vizioso delle procedure di infrazione in cui molto spesso (*Segue* MAZZONI). Forse questo disegno di legge giunge in sede di approvazione definitiva addirittura troppo tardi, se si considerano, oltre alle già citate sanzioni in caso di mancato ottemperamento all'adeguamento alla normativa europea, soprattutto i benefici derivanti da una sempre maggiore conformità legislativa interna a quella quella dell'Unione. Recepire gli indirizzi sovranazionali e conformarsi alle direttive europee rappresenta, infatti, anche un'opportunità di non poco conto per la crescita in termini economici del nostro Paese. La possibilità di agevolare la nostra partecipazione alla tanto auspicata nuova politica di investimenti europea rappresenta un'occasione importante che non deve essere sprecata per strumentalizzazioni politiche o irresponsabili prove di forza tra maggioranza e opposizioni. Anzi, dalle Aule parlamentari dovrebbe giungere un forte incentivo comune per far sì che l'Italia possa essere sempre più determinante in Europa, anche partecipando in maniera sempre più attiva alla stesura e alla formazione della normativa dell'Unione europea, che devono essere figlie di una politica comune, concordata e portata avanti con determinazione. Dobbiamo partecipare con sempre maggiore incisività alle decisioni quadro e perché ciò avvenga è necessaria la preliminare attuazione delle norme di indirizzo contenute nelle direttive che vanno recepite, anche se non supinamente, e inserite nella nostra legislazione. Fatta questa il provvedimento che stiamo discutendo dovrebbe consentire l'archiviazione di tre procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e superare altre contestazioni già mosse al nostro Paese, così da evitare l'apertura formale di altre procedure. Serve, però, anche un impegno maggiore del Governo per far valere con determinazione le nostre esigenze di carattere economico, in modo da rivitalizzare il nostro tessuto produttivo per metterci alla pari con i Paesi europei più forti e per sollecitare con maggiore determinazione un'Europa realmente unita con politiche comuni basate su scelte condivise. Il raggiungimento di questo obiettivo, le cui conseguenze impattano direttamente sulla vita dei cittadini, ci deve vedere protagonisti nelle grandi decisioni che l'Europa è chiamata a prendere. Non dobbiamo subirle, come spesso purtroppo è accaduto, ma proporle. Per fare ciò è però necessario procedere all'armonizzazione delle normative interne a quelle sovranazionali, così da garantire nell'immediato, ma con un'ottica di lungo periodo, un'interconnessione del tessuto economico e sociale a livello europeo talmente sviluppata da rendere talmente sviluppata da rendere il processo verso un'Europa politica un passaggio obbligato. Per questi motivi avrei dovuto dichiarare il voto favorevole del Gruppo ALA - Scelta Civica a questa legge di delegazione europea 2017. quantomeno discutibile. Parlo dell'articolo 5, che contiene una norma di due righe che modifica la legge Mancino e che creerà gravissimi problemi nella sua interpretazione e applicazione. Introdurre, infatti, la minimizzazione storica dei crimini commessi contro l'umanità, così come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, come fattispecie di reato, è un passo, a nostro avviso, molto pericoloso Voglio essere chiaro: non c'è alcun dubbio che, facendo riferimento all'Olocausto e alla sua unicità, il negazionismo non può trovare un solo sostenitore e che siamo di fronte al più grande crimine compiuto nella storia dell'umanità, ma la verità storica - lo dicono gli storici e non io - non è materia di competenza dei tribunali. Inoltre, quando si parla di minimizzazione, si definisce una categoria assolutamente indeterminata e difficilmente determinabile. Ciò è tanto più grave perché qui si determinano anni di carcere e non una semplice multa. Questa legislatura si è distinta per applicare e inventare fattispecie di reato molto vaghe che non fanno lavorare bene i giudici e che sono un grave peccato del legislatore. Per tale ragione, essendo stato approvato l'articolo 5, il nostro Gruppo non può votare favorevolmente al provvedimento e si asterrà. Signor Presidente, in questo giorno è stata inferta una grave ferita alla democrazia. La legge elettorale che ci si appresta a votare alla Camera impedisce agli elettori di scegliere i parlamentari. La fiducia su questa legge elettorale, imposta dal Governo su una legge squisitamente parlamentare, impedisce ai parlamentari di discutere la legge più importante per la democrazia del Paese. Tutto ciò viene fatto contro una delle componenti della maggioranza: si sceglie scientemente di estromettere Articolo 1-MDP da questa maggioranza. La legge europea che ci apprestiamo a votare è un atto importante dell'azione del Governo e la sua maggioranza ha il dovere di sostenerla. Lo faccia. Per quanto ci riguarda, noi ci asterremo.

La legge europea, dunque, è non solo uno strumento tecnico utile per ridurre il numero di contenziosi che le istituzioni comunitarie hanno sollevato nei confronti dell'Italia, ma un vero e proprio investimento politico del nostro Paese nel percorso di avvicinamento della normativa nazionale a quella europea. una scelta che riteniamo strategica e qualificante e che abbiamo rafforzato e ribadito costantemente in questa legislatura. Infatti, questa determinazione ha consentito, in poco più di tre anni, di dimezzare il numero di procedure di infrazione e di fare dell'Italia il Paese più virtuoso nella gestione dei casi di contenzioso comunitario. del provvedimento in esame chiuderemo altre tre procedure di infrazione e definiremo altri sette casi EU Pilot. Sappiamo perfettamente che l'Italia rimane uno dei Paesi con una situazione di contenzioso con l'Unione europea abbastanza critica, ma è altrettanto evidente come il lavoro costante degli ultimi anni ci abbia portato a raggiungere oggi il minimo storico di 65 procedure aperte. Si tratta di un obiettivo ottenuto grazie a una duplice attenzione: da un lato, la capacità di intervenire con rapidità in fase sia di contenzioso, che di prevenzione e, dall'altro lato, l'accresciuta compatibilità della legislazione italiana con quella comunitaria, a testimonianza di una maggiore consapevolezza dell'impatto positivo che le politiche europee possono avere anche nel nostro Paese. Nel 2016, rispetto al numero di nuove procedure di contenzioso aperto, l'Italia ha fatto meglio di Germania e Francia e nel medesimo anno questo percorso virtuoso si è tradotto in un'economia di oltre 180 milioni di euro. oltre alle evidenti convenienze economiche, questo risultato testimonia concretamente come per Governo e Parlamento il tema della costruzione europea non sia un vessillo da utilizzare solo nel momento del bisogno, quanto - piuttosto - un convincimento profondo circa la necessità di tradurre i valori e i principi comunitari in scelte che accelerino l'integrazione e rafforzino le tutele dei cittadini europei. Con la legge europea mettiamo dunque i cittadini e le imprese italiane nelle condizioni di poter beneficiare, al pari degli altri cittadini europei, dei maggiori diritti e delle migliori garanzie che le normative comunitarie prevedono, in virtù della capacità dell'Europa di poter rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative delle persone.

Oltretutto, con l'approvazione del provvedimento si amplierà il campo di applicazione dell'aggravante di negazionismo e si interverrà sulla disciplina dell'indennizzo alle vittime di reati intenzionali e violenti, estendendone l'ambito di applicazione. Altra norma rilevante è quella in materia di *roaming*. Infatti, il 15 giugno di quest'anno il Parlamento europeo ha rimosso l'ultimo ostacolo all'abolizione dei costi di *roaming*, consentendo a tutti i cittadini europei di utilizzare telefonini, *smartphone* e *tablet* senza costi aggiuntivi mentre si viaggia in Europa. Per rendere pienamente efficace questa novità era però necessario intervenire nell'ordinamento nazionale, introducendo le sanzioni per la violazione delle disposizioni europee ed è ciò che abbiamo fatto. Il testo del disegno di legge in esame interviene anche in materia di commercio elettronico, per rafforzare le responsabilità per gli operatori che commettono illeciti; introduce rilevanti disposizioni in materia fiscale, consentendo ai cittadini e alle imprese italiane di usufruire delle medesime possibilità di tutti gli altri cittadini europei; novella la normativa nazionale in materia di aiuti di Stato ed energia. Dopo un lungo negoziato, abbiamo infatti finalmente adottato gli indirizzi comunitari sulle aziende energivore e, contemporaneamente, sfruttando i risparmi della componente A3, ridurremo ridurremo i costi delle bollette per le famiglie e le imprese non energivore. Si tratta di una previsione di grande equità che aiuta le imprese e, quindi, l'occupazione e le famiglie. diritti dei cittadini europei, mercato unico digitale e politiche fiscali omogenee: sono molti gli aspetti che contribuiscono a rendere concreto il senso di cittadinanza europea e con il provvedimento in esame avviciniamo ancora di più l'Italia all'Europa. però anche consapevoli che il terreno della sfida non è semplicemente quello relativo ai singoli interventi. Sullo sfondo pesa la crisi profonda che l'Unione europea sta attraversando. Per avvicinarci all'Europa dobbiamo saper coniugare la strada percorsa finora, costruita su conquiste quotidiane di cittadinanza, con una strada nuova, capace di rinnovare un vero e proprio patto sociale europeo. I Governi nazionali e le forze politiche troppo spesso parlano solo al proprio pubblico, senza pensare a un futuro in comune, cavalcando il sentimento di insicurezza e sfiducia, spesso senza saper guardare oltre la propria frontiera. Non possiamo avvantaggiarci di essere europei per risparmiare sulle tariffe telefoniche per navigare in Internet dall'estero, ma dimenticare questo comune destino quando si tratti di pianificare una condivisione ordinata e sociale dell'emergenza migranti o quando si chiedano maggiori risorse per politiche di protezione sociale. Per questa ragione, con la stessa determinazione con cui in questi anni abbiamo lavorato per avvicinare gli italiani all'Europa, riteniamo fondamentale proseguire nello sforzo di avvicinare l'Europa agli italiani. Per queste ragioni, solo attraverso una condivisa e rinnovata strategia europea si può sperare di rilanciare il processo di integrazione e con il disegno di legge in esame andiamo esattamente in questa direzione. Esprimo pertanto, a nome del Gruppo di Alternativa Popolare, il voto favorevole al presente provvedimento e al tempo stesso, come Gruppo, ribadiamo il nostro impegno affinché l'Europa torni ad essere strumento reale e concreto di coesione e di pace, in grado di creare una nuova ragione sociale comune. Voteremo a favore guardando all'interesse nazionale e con la responsabilità piena di una forza politica convintamente europeista, che non intende mai cedere a facili slogan e populismi, ma continua con serietà a percorrere la strada dell'integrazione europea. la legge europea rappresenta uno strumento particolarmente qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento degli obblighi e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione europea. Con il testo oggi al nostro esame siamo chiamati, come di consueto, ad adeguare siamo chiamati, come di consueto, ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In linea generale, quindi, periodicamente ci occupiamo di norme tese a prevenire l'apertura di procedure di infrazione o a chiuderle, sanando situazioni che, in base ai pronunciamenti degli organi giurisdizionali europei o ai richiami della stessa Commissione europea, non sarebbero in armonia con la legislazione europea. La *vexata quaestio* sul negazionismo ne è un esempio anche se è difficile seguire l'Europa su tale materia senza fare torto alle coscienze degli uomini liberi e delle donne libere. modo non possiamo sottacere gli sforzi italiani per rientrare nei canoni delle infrazioni palesi: qui i risultati sono sotto gli occhi di tutti. All'interno di questo disegno di legge troviamo numerosi importanti argomenti: si spazia dalla giustizia alla sicurezza e si finisce con il lavoro, l'ambiente, insomma si fa fatica a guardare la natura di questo provvedimento. Ritengo che l'Europa non possa essere solo questo: si prendono tante piccole decisioni, ma non si riesce a far fare un passo in avanti affinché il nostro Paese dia un contributo al rafforzamento della sua posizione in seno al consesso dell'Unione europea. Le finalità del presente sono di ridurre o addirittura di rimuovere i casi di contrasto normativo tra il nostro ordinamento e quello europeo, ma nei fatti il disegno di legge oggi alla nostra attenzione tiene conto in maniera marginale delle esigenze dell'interesse nazionale, dei nostri cittadini e delle imprese, sempre più nei morsi della crisi del nostro tessuto sociale ed economico in affanno. Non si affrontano le gravi emergenze, il protrarsi di una grave crisi occupazionale, dei giovani in bilico tra disperazione o condanna al precariato. Non vi è solo la grande emergenza dell'immigrazione, di cui non si può non parlare per il risvolto umano, ma anche per la difficoltà dell'Europa e dei Paesi europei ad avere una capacità effettiva di accoglienza e di integrazione. Da gennaio di quest'anno sono più di 100.000 gli immigrati che sono sbarcati sulle nostre coste, un esodo di massa di gente che fugge da guerre e da gravi situazioni economiche e che a fatica riusciamo a gestire, mentre l'Europa sta a guardare. Sul lavoro deteniamo purtroppo il *record* dei giovani che non studiano, che non lavorano e che non cercano più un'occupazione. I dati della Commissione ci dicono che circa il 20 per cento dei nostri giovani si trova in questa condizione, mentre la media europea si attesta cento. Il nostro Paese ha un livello di tassazione diventato insopportabile per le famiglie, le imprese ed i professionisti e che andrebbe rivisto al più presto. C'è bisogno di una profonda riflessione sul futuro del progetto europeo, tornare ad essere protagonisti e dimostrare ai nostri cittadini che l'Unione europea rappresenta una risorsa per lo sviluppo, necessita di unione autentica e di cooperazione vera. L'Unione europea non può essere solamente quell'entità burocratica capace di vincolarci e di ostacolarci, intervenendo a gamba tesa sulle tradizioni e sulle culture locali, addirittura sulle biotipicità e sui costumi. Un appuntamento che potremmo cogliere per svolgere un ruolo propulsivo e propositivo importante sarà quello di fine anno Ritengo che il compito di un Governo sia difendere gli interessi dei propri cittadini e delle imprese nazionali. Non si deve avere un atteggiamento rinunciatario nei confronti della Commissione europea; bisogna andare a negoziare, ogni qualvolta ci siano procedure di infrazione che mettono in ballo gli interessi del nostro Paese. Certamente noi dobbiamo ottemperare ai nostri obblighi, e da qui l'approvazione di questa legge, ma bene anche la critica costruttiva alla situazione generale. Le nostre posizioni critiche non sono indirizzate ad aver meno Europa, ma a realizzare più Europa, nel rispetto delle specificità e delle prerogative delle Nazioni, perché solo più Europa può salvare l'Europa stessa e i singoli Stati che ritengono di salvarsi ricorrendo al fai da te. Per queste e per molte altre considerazioni che sarebbero da muovere, mi sento

Signor Presidente, proprio alcuni giorni fa la Commissione europea ha adottato le sue decisioni in materia di procedure di infrazione. Per quanto riguarda l'Italia, il numero delle procedure a carico del nostro Paese è lievemente sceso ma rimane a quota 64, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. Si rileva come la legge in discussione presenti soltanto 29 disposizioni più l'articolo relativo all'invarianza finanziaria. Come sempre, la materia ambientale la fa da padrona con ben 16 procedure ancora aperte e su materie per nulla irrilevanti: mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti, convalida dei dati e ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria, riduzione dell'utilizzo di buste di plastica in materiale leggero, violazione della direttiva habitat per la mancata designazione delle zone speciali di conservazione e adozione delle misure di conservazione, l'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto, il superamento dei valori limite di PM10 in Italia, l'immancabile trattamento delle acque reflue urbane, l'ILVA di Taranto, le discariche e l'emergenza rifiuti in Campania, poi passare ad altri settori che vedono infrazioni su materie come la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi o la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e la xylella fastidiosa. Ci si chiede, allora, signor Presidente, quale sia la logica che spinge il Governo ad intervenire su alcuni fronti lasciando altri del tutto scoperti. Quale sia il criterio di urgenza nell'intervenire su alcuni temi, ignorandone altri. La sensazione che si ha, purtroppo, è sempre quella di un utilizzo improprio dei vincoli e degli obblighi che ci impone l'appartenenza ad un'istituzione sovranazionale, vincoli che diventano un comodo scarico di responsabilità qualora le misure intraprese risultino impopolari, per cui alcune strade vengono presentate come obblighi europei e non come scelte di politica del Governo. vincoli, però, possono essere tranquillamente ignorati quando invece sono rivolti a tutelare i cittadini, a tentare di imporre regole che consentano alle persone di vivere in una società più salubre e più equa.

Ecco, quindi, che un vincolo dell'Unione europea posto a tutela dei consumatori e della concorrenza fra aziende che volessero investire nel campo del cosiddetto viene bellamente ignorato in sede di discussione sia in Commissione sia in Aula. Come Sinistra Italiana, avevamo presentato emendamenti e degli ordini del giorno tesi proprio a legiferare per porre fine a questa pratica scorretta a danno dei consumatori. Eppure, signor Presente, si va anche al di là:

come è successo in questo disegno di legge, norme in palese contrasto con la legislazione europea. È questo il caso, ad esempio, dell'articolo 2 e della famosa questione riguardante il diritto d'autore. Con l'articolo 2 si dà all'Agcom, l'autorità governativa *per* le garanzie nelle *comunicazioni*, il potere di erogare misure cautelari nel campo della salvaguardia al diritto d'autore.

2004/48 - quella che si dice di voler recepire all'articolo 2 - prevede che gli Stati membri assicurino che le competenti autorità giudiziarie siano i soggetti preposti a prendere tali misure cautelari nei confronti di soggetti soggetti imputati della violazione del diritto d'autore. Quindi, ecco che, su una materia che l'Europa stessa ci dice che giustamente deve essere messa in mano all'autorità giudiziaria, questo Governo, con un articolo ancora una volta di dubbia legalità,

Una parte autorevole della dottrina qualifica l'Agcom - pensate, colleghi - come autorità semi-indipendente. Infatti, un'autorità amministrativa indipendente è tale se non è subordinata né gerarchicamente né politicamente ai Ministeri, e non è questo il caso dell'Agcom. Quindi, stiamo dando - badate bene, colleghi, signor Presidente - poteri cautelari propri della magistratura a un'autorità semi-indipendente, quindi nelle mani del Governo, che avrà pertanto il potere di censurare Internet qualora rilevi, essa agenzia, che si possa essere verificata una violazione del diritto d'autore. Signor Presidente, a me questo articolo suona poco democratico davvero; poi, naturalmente, ai posteri l'ardua sentenza. Questo è anche il caso, come abbiamo visto poco fa, proprio in occasione di un mio intervento sull'articolo 24,

che il periodo di conservazione delle telefonate sia di due anni e quello delle telefonate non risposte soltanto di trenta giorni - pensate - mentre il traffico Internet soltanto di un anno. Ecco che il Governo, con un autentico colpo di mano illiberale, aumenta in modo indiscriminato questo periodo a sei anni, violando addirittura la direttiva europea che si vuole recepire in quanto la stessa direttiva parla di misure di contrasto al terrorismo e applicazione di sanzioni per il contrasto al fenomeno dei *foreign fighter* mentre il Governo aumenta questa *data retention* e dà la possibilità di mettere mano a questa schedatura indiscriminata degli utenti anche per tutta un'altra serie di reati che non hanno a che fare con il terrorismo internazionale. Dunque, signor Presidente, com'è possibile quindi che, quando si tratta di rispettare le norme in materia di rifiuti, di inquinamento dell'aria e dell'acqua, di trattamento delle acque, di agricoltura, di quote latte, di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (come abbiamo visto), di condizioni di accoglienza per i richiedenti asilo e di tutti quegli altri fondamenti e aspetti sistematicamente violati dalla nostra normativa (come ci ricordano le 64 procedure di infrazione ancora aperte), il Parlamento e il Governo rispondono con un'alzata di spalle e un arrivederci all'anno prossimo, se non quando addirittura con uno stravolgimento dei vincoli stessi, e invece, quando si tratta di mettere in discussione vincoli a sistemi economici profondamente lesivi dei cittadini, le mani risultano improvvisamente legate dall'Europa? Lo vedremo, perché, entro fine anno, i Parlamenti nazionali dovrebbero discutere e decidere il destino del *fiscal compact*. Fermiamoci finché siamo in tempo e imponiamo invece all'Europa misure più eque e di ampio respiro e non vessatorie della libertà di cittadini, come ad esempio un piano di investimenti pubblici, destinato a interventi medio-piccoli e verdi, il congelamento di accordi di libero scambio, come il CETA e il TTIP, anche questi in palese violazione dei diritti dei consumatori, l'introduzione di *tobin tax* e *web tax*. Soprattutto però le istituzioni dovrebbero, senza ritardi e giustificazioni, rispettare la legislazione europea quando essa è rivolta ai cittadini, italiani, europei o di qualsiasi parte del mondo. Per questo motivo, signor Presidente, noi componente Sinistra Italiana del Gruppo Misto ci asterremo dal voto di questo disegno di Signor Presidente, anche noi vorremmo stigmatizzare quanto sta succedendo alla Camera dei deputati, con l'esame e l'approvazione della legge elettorale. Non lo vogliamo stigmatizzare perché siamo esclusi dalla maggioranza (per noi questo è un onore), ma perché a nostro avviso si stanno escludendo i cittadini dalle elezioni *(Applausi dal toglie loro la possibilità di scegliere e di non vedere disperso il proprio voto. Ecco perché noi ci sentiamo di stigmatizzare questo colpo inferto alla democrazia. Detto questo, tornerò

65 procedure, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 10 per mancato recepimento di direttive. E questo la dice lunga sul nostro Paese. Guardate, tra le ultime procedure per infrazione aperte c'è la n. 2017/2090, che riguarda la compatibilità del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, il correttivo appalti; e stiamo andando in infrazione.

quella sull'osservanza della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Evidentemente non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare, contrariamente a quanto diceva oggi il sottosegretario Gozi, che diceva che siamo stati bravi perché abbiamo dimezzato il contenzioso europeo. A me pare non ci sia alcunché di cui andare fieri, perché in realtà, come abbiamo visto, il contenzioso è ancora corposo. Questo sicuramente perché in Italia si verifica il fenomeno del *gold plating*, ovvero una sovraregolamentazione che porta a procedure di infrazione per errato recepimento. Una bulimia normativa che sta portando a approvare provvedimenti su provvedimenti perdendo di vista il bene comune. E quando occorre adeguarsi alla normativa non si trova più il bandolo della matassa, con i risultati che ho appena detto, ad esempio in merito al correttivo degli appalti 2017. Oppure perché recepiamo le direttive con un occhio che guarda l'Unione europea e un occhio che, invece, guarda ad interessi del tutto italiani. Un caso è proprio quello della SIAE,

dal 2014 questa situazione anomala, presentando emendamenti e ordini del giorno all'interno di vari provvedimenti, tra i quali anche la legge europea votata mesi fa. mesi fa. Finalmente, mesi fa il Governo si è deciso ad approvare un ordine del giorno che lo impegna, nella imminente legge di bilancio, a sanare una volta per tutte questa situazione che è scandalosa.

questo organismo di garanzia ha la possibilità di oscurare i siti Internet attenzionati per supposte violazioni del diritto d'autore e ha la possibilità di oscurarli in via precauzionale, in attesa che a decidere se effettivamente questa violazione vi sia stata oppure no sia l'organo preposto dalla legge, ovvero la magistratura. Con questo emendamentino, invece, l'Agcom avrà anche la facoltà di emanare provvedimenti in via Quindi, si crea qui una confusione tra le prerogative di una autorità giudiziaria e le prerogative di un organo di garanzia; questo mi pare molto grave da parte di un Parlamento e di una forza politica di maggioranza.

le decisioni prese dall'Agcom? Alla Agcom stessa! E chi deciderà le modalità con cui sarà disciplinato questo reclamo? L'Agcom stessa! Perché voi siete capaci di fare

approvare un nostro emendamento che si basava sul principio europeo di precauzionalità in materia di ambiente e di salute pubblica. Non avete poi voluto approvare un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che richiamava l'attenzione

potrebbe essere dannoso per la salute ambientale e, quindi, anche per la salute delle persone, ma voi non avete voluto ascoltarci neanche su questo. Per tutte queste ragioni, il Movimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione sulla legge europea. E chissà che la legge europea non sia occasione per dimostrare quanto abbiamo fatto bene a votare no al *referendum* costituzionale e a mantenere in vita questo ramo del Parlamento. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori Ministri presenti, è con piacere che svolgo la dichiarazione di voto sulla legge europea. Oggi si è infranto il patto che esisteva tra Camera e Senato, sulla base del quale la competenza della legge

*misunderstanding* tra il Senato e il Sottosegretario o comunque tra Parlamento e Governo, due emendamenti che potevano essere trasformati in ordini del giorno, senza alcun alcun mutamento dello spirito della legge, sono stati votati e hanno prodotto l'esito che tutti noi conosciamo. Ciò fa sì che il anziché essere approvato in via definitiva, debba ritornare alla Camera per un ulteriore passaggio parlamentare. Questo comporterà

e non avremo comunque una legge particolarmente modificata nei suoi contenuti, se non per due non rilevanti, ma comunque importanti, emendamenti: uno sull'etichettatura, che resta

Sottosegretario, perché una forza che vi sostiene e vi ha sempre sostenuti fino a oggi dichiara che si asterrà nel voto finale sul disegno di legge. legge. Evidentemente, non è la condivisione verso i nostri emendamenti che ha spinto a questo atteggiamento la forza di cui sto parlando, ma è certamente

all'Europa, risolvendo il problema dei migranti con risorse proprie. Avremmo voluto che ci fosse all'interno di questa legge anche un qualcosa che riguardasse la direttiva Bolkenstein. Avremmo voluto ancora di più che ci fosse qualcosa all'interno della legge che riguardasse i debiti della pubblica amministrazione verso le 20.000

e tranquilla, senza particolari increspature in Commissione, dopo essere stato approvato da molti Gruppi parlamentari anche alla Camera dei deputati. È quindi un po' con sorpresa che oggi vediamo tutta questa questa agitazione intorno ad alcune norme che non avevano sollevato alcuna perplessità nel momento in cui c'era la possibilità di approfondire nel merito, nelle sedi proprie.

rimane il sospetto che alcune differenziazioni che oggi si sono manifestate abbiano poco a che vedere con il merito del provvedimento, ma riguardino altre vicende, che si stanno svolgendo in altri luoghi. Signor Presidente, vorrei l'Europa è un ecosistema fragile, una realtà di cui dobbiamo farci carico e sentirci responsabili tutti insieme. Non possiamo pensare che sia una realtà irreversibile.

Certo, il nostro spirito europeo ci porta a fare il tifo per chi oggi vuole costruire l'Unione europea e non per chi la vuole distruggere, per chi la vuole rafforzare e non per chi la vuole rendere Credo che in questi giorni abbiamo avuto di fronte atteggiamenti, a tratti, di irresponsabilità di coloro che non hanno percepito con chiarezza quale sia il beneficio che l'Europa ha portato al nostro Continente in tutti questi anni

voglio anche dire che non è necessariamente un fatto negativo che vi siano procedure di infrazione, perché non è che ogni qual volta l'Europa ci chiede di modificare la nostra legislazione dobbiamo immediatamente accorrere e, allo schioccare di dita, precipitarci a farlo. Noi, in certi casi, facciamo bene a resistere e a mantenere un atteggiamento di contraddittorio in un contenzioso per sostenere le nostre ragioni e quindi è giusto che ci siano anche delle procedure che pendono, perché questa è la dimostrazione della nostra capacità di far valere il buon diritto, le scelte politiche, le scelte legislative e le scelte amministrative del nostro Paese. Certo, questo tipo di atteggiamento deve essere portato avanti con lungimiranza ed attenzione. Sono convinto che l'Italia sia migliorata e sia oggi un Paese migliore grazie alle politiche europee e grazie anche al contributo contributo di scelte condivise con altri Paesi, che hanno portato a rendere il nostro un Paese più moderno ed efficiente. Dobbiamo anche renderci conto che c'è un numero importante di procedure d'infrazione legate non alle scelte legislative, bensì ad

locali sugli atti e sui passi da intraprendere per ridurre il contenzioso e mettere il nostro Paese al passo con l'Unione europea. Vorrei avviarmi alla conclusione di questo mio intervento, signor Presidente, ricordando che ricordando che oggi parliamo di un provvedimento che riguarda l'aspetto patologico, che riguarda cioè l'Europa dal punto di vista delle infrazioni, ma dobbiamo sempre di più essere consapevoli che il nostro ruolo all'interno dell'Unione europea sarà forte non soltanto quando riusciremo a ridurre il numero di infrazioni, cosa che sicuramente di per sé aumenterà la nostra credibilità, ma nel momento in cui saremo in grado di portare avanti la voce dell'Italia, di farla sentire e di far pesare la visione italiana nel dibattito europeo. Oggi assistiamo ad una

nella prima tornata elettorale e poi, grazie al ballottaggio, con una percentuale molto più alta, riesca ad avere un ruolo di *leadership* all'interno dell'Unione europea. Economist», provocatoriamente, mette proprio Macron sotto i riflettori ed Angela Merkel in secondo piano. Noi siamo vincolati dalle decisioni prese dalla nostra Corte costituzionale, che nella sua suprema saggezza ha deciso che il ballottaggio non è fatto per gli italiani,

legato al proporzionale anziché al maggioritario - ma credo che sarà comunque necessario avere una forte coesione ed una forte capacità di comunità d'intenti.

mi auguro che la Camera possa rapidamente approvare le modifiche che oggi abbiamo apportato al disegno di legge e soprattutto si possa scongiurare quello che per me è il rischio peggiore, e cioè che vadano persi dei finanziamenti che erano stati previsti per la Sardegna, in particolare per la regione del Sulcis, che dovevano essere destinati entro la fine dell'anno pena la perdita dell'intero finanziamento. a perdere questi finanziamenti europei per i sardi, sarebbe uno smacco non soltanto per la credibilità italiana e per l'avanzamento del nostro percorso in Europa, ma sarebbe anche una grave perdita per dei nostri cittadini, che credo non se lo meritino. Mi auguro pertanto che i nostri colleghi alla Camera riescano a procedere rapidamente. Detto ciò, non posso che concludere il mio discorso dichiarando il voto favorevole del Partito Democratico a questo disegno di legge.